L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un senatore Segretario. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento, ciascun senatore scriverà sulla propria scheda un solo nominativo. Risulterà eletto il senatore che otterrà il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età. Per garantire il più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, dinanzi al banco della Presidenza sono state predisposte due cabine. I colleghi senatori, immediatamente prima dell'ingresso in cabina, riceveranno dagli assistenti parlamentari la scheda che, dopo il voto, depositeranno nell'apposita urna all'uscita della cabina stessa. La chiama sarà svolta in ordine alfabetico. Dichiaro pertanto aperta la votazione e invito il senatore Segretario a procedere all'appello.

Invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede e al computo dei voti nell'adiacente Sala Pannini.

Signora Presidente, il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*. È un testo che è già stato approvato dalla Camera dei deputati e si compone di tre articoli. Durante l'esame da parte della Camera dei deputati non sono stati approvati emendamenti, ma solo modifiche di *drafting* riguardanti il coordinamento formale del testo. L'articolo 1 del decreto-legge è diretto a prorogare, salve minime correzioni, l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento con riferimento all'esecuzione delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e di vaglio dell'ammissibilità dei quesiti referendari. Infatti, come indicato dal preambolo del decreto-legge, in attesa della piena operatività della piattaforma digitale, è necessario rafforzare gli Uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che, in forza dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, devono essere svolte dal 30 settembre al 31 ottobre, in attesa prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Considerando la possibilità di raccogliere le firme in modalità digitali, per quanto riguarda la sottoscrizione dei *referendum* introdotta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, senza che nel frattempo sia divenuta operativa la detta piattaforma digitale prevista dalla stessa legge, si propongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta firme, ma con scarse garanzie in termini di autenticità e soprattutto senza semplificare le attività di verifica. Per consentire la piena operatività dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, il decreto-legge dispone quindi un temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate dopo il 31 ottobre 2021. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che l'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione si avvalga di ulteriore personale della segreteria della medesima Corte, nel numero massimo di 28 unità, anche appartenenti all'area assistenti, già inquadrato nel comparto Ministeri seconda fascia, fascia economica da F4 a F6. Tale disposizione costituisce una deroga all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, che prevede che per le operazioni di verifica l'Ufficio centrale per il referendum si debba avvalere del personale della segreteria con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Per le medesime finalità, il comma 2 dell'articolo 1 consente al primo Presidente della Corte di cassazione di avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in in servizio presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui: 40 unità destinate alla funzione di verifica e conteggio delle sottoscrizioni (appartenenti all'area assistenti già inquadrati nel comparto Ministeri seconda fascia, fascia economica da F4 a F6); 60 unità con mansioni esecutive di supporto, quale l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, (appartenenti all'area assistenti già inquadrato nel comparto Misteri, seconda area, fascia economica da F1 a F3). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, all'acquisizione di disponibilità all'assegnazione all'Ufficio centrale per il referendum, si provvede mediante interpello per soli titoli indetto dall'amministrazione giudiziaria su richiesta del primo Presidente della Corte di cassazione. Come previsto dal successivo comma 4, si prevede che possano partecipare all'interpello i dipendenti di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbiano maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza. Il comma 5 dell'articolo 1, oltre a disporre in materia di retribuzione del personale aggiuntivo assegnato a seguito dell'interpello, stabilisce che tale personale sia responsabile presso l'Ufficio centrale delle operazioni effettuate. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, ai sensi delle quali il primo Presidente dispone sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario; inoltre, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 199 del 1978 il primo Presidente della Corte di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di referendum, con proprio decreto e in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il referendum altri magistrati della Corte. L'articolo 2 del decreto-legge introduce invece la disciplina della piattaforma telematica per il referendum prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la raccolta delle firme degli elettori necessari per il referendum e le iniziative legislative popolari. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, introducendo all'articolo 1 della citata legge 2020, il nuovo comma 342-bis, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024 la titolarità della piattaforma sia attribuita al Ministero della giustizia e che, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la realizzazione della piattaforma sia iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero della giustizia. L'articolo 3 dispone, infine, in merito all'entrata in vigore del decreto-legge. [**Presidenza

comparto, quello appunto della struttura dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di cassazione, che ha il merito di consentire, attraverso attraverso l'uso di un istituto giuridico, quale appunto il *referendum*, l'esercizio della democrazia diretta da parte dei cittadini e di farlo in particolar modo su argomenti sui quali spesso anche la politica non ha la forza o il coraggio di intervenire in maniera decisa. Si tratta nella storia referendaria di temi che a volte toccano anche l'etica e che quindi, comprensibilmente, sono oggetto di discussione anche nelle sedi istituzionali, con divisioni che non rispettano solitamente le divisioni politiche, ma vanno a coinvolgere anche gli aspetti più personali di ognuno di noi. Pertanto, non possiamo che dirci d'accordo con la finalità che questo disegno di legge vuole perseguire, ovvero quella di risolvere un problema organizzativo per il supporto necessario Corte di cassazione ad assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che abbiamo avuto modo, anche da ultimo, di seguire attraverso le attività sui *referendum* della giustizia, fortemente voluti dalla Lega, che - è vero - hanno magari visto partecipare solo una percentuale del corpo elettorale, non raggiungendo quel limite oltre il quale avremmo ottenuto la validità dei quesiti, ma permettono ai cittadini di potersi esprimere contro o a favore

Signor Presidente, voglio cominciare questa mia breve dichiarazione di voto facendo i complimenti al Governo per aver finalmente emanato, dopo più di un anno di lavoro, il primo decreto-legge che rispetta l'articolo 77 della Costituzione. *(Applausi)*. Congratulazioni, è nato il bebè: finalmente abbiamo un decreto-legge che viene adottato per ragioni di necessità ed urgenza. Speriamo di non vederne soltanto uno ogni però è chiaro che in questo caso, se la Corte di cassazione non ce la fa a valutare ed esaminare la documentazione che giace presso di essa credo - proposte referendarie che sono pendenti, è giusto che il Governo ne prenda atto e urgentemente distacchi del personale di altre pubbliche amministrazioni presso la Corte di cassazione. ovviamente di un pannicello caldo, perché se noi comandiamo personale da altre pubbliche amministrazioni alla Corte di cassazione, vuol dire che andiamo a dare una mano alla Corte di cassazione e togliamo personale alle amministrazioni di provenienza e quindi probabilmente creiamo dei problemi mentre ne risolviamo degli altri. una visione strutturale delle piante organiche sarebbe utile. Però, la democrazia diretta, quella referendaria, è importante, non quella che vuole abolire il Parlamento e sostituirlo con dei portavoce o con dei *click*, ma quella prevista dalla Costituzione va preservata e quindi è bene che si Il secondo punto di questo provvedimento riguarda la famosa piattaforma che dovrebbe andare a sostenere

capillare e anche dei fondi necessari a coprire le spese per l'organizzazione dei banchetti e l'autenticazione delle firme poteva effettivamente portare il *referendum* e la raccolta delle firme a compimento. È chiaro che la domanda che nasceva spontanea, posto l'avanzamento tecnologico, è perché l'autenticazione delle firme non potesse avvenire tramite l'utilizzazione dello Spid. Infatti, grazie a una modifica normativa che risale soltanto a pochi anni fa,

ci ha insegnato che è vero il contrario. Le firme sono state raccolte per *referendum* importanti, *referendum* che purtroppo, come quello sulla legalizzazione della *cannabis*, hanno trovato un ostacolo nella valutazione della Corte costituzionale, della quale naturalmente rispettiamo esiti, esiti, giudizi, decisioni, anche se poi non sempre siamo obbligati a condividerli. Insomma, la facoltà di dare la propria firma con lo Spid non è stata fatta oggetto di abusi. Purtroppo, quello che succede è che quella piattaforma, che dovrebbe essere pubblica e che la legge prevede, a distanza di più di due anni non è stata ancora predisposta. Pertanto, negli unici casi nei quali si è utilizzata la raccolta firme con lo Spid, sono stati i comitati organizzatori a dover organizzare delle piattaforme private,

intuisco sarà responsabile di questo processo. Gli saremo vicini per verificare che tutto questo avvenga, perché è ovvio e giusto che tutto questo possa accadere. Tra l'altro, segnalo ai colleghi senatori e senatrici che alla Camera sono stati presentati ordini del giorno affinché questo strumento possa essere utilizzato anche per le leggi di iniziativa popolare. Penso che sia un dato molto importante, perché sappiamo che questo è un istituto molto rilevante della nostra Costituzione, che purtroppo raramente (possiamo dire quasi mai) riesce a partorire i frutti che erano nella mente dei nostri costituenti. A me non resta che annunciare il voto favorevole del Gruppo di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe a questo provvedimento. Auspichiamo, naturalmente, che passi con un largo consenso, ma trattandosi decreto-legge, come tutti sappiamo, le norme sono già in vigore. Bisogna convertirlo e io penso che non ci sia alcuna ragione per non farlo subito. Quindi, oltre ad annunciare il nostro voto favorevole, auspico che l'intero Senato voglia votare favorevolmente e che finalmente questo provvedimento entri a pieno titolo nel nostro ordinamento. intervengo solo per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo. Io credo che tutti gli strumenti che peraltro vengono previsti in in questa conversione in legge del decreto-legge, che in qualche modo rendono più semplice la possibilità di accedere agli strumenti di democrazia diretta, vadano con forza sostenuti. Quindi, mi rallegro e considero positivo il fatto che da oggi, nel nostro Paese, sia più facile poter accedere all'indizione del *referendum*. Credo che sia giusta la sottolineatura che è stata fatta adesso dal senatore Scalfarotto: è altrettanto giusto e altrettanto importante che questa cosa riguardi anche le leggi di iniziativa popolare,

che poi si passi dalle parole ai fatti e che effettivamente per il *referendum*, ma anche per le leggi di iniziativa popolare, si consenta realmente ai cittadini che firmano di essere protagonisti di una discussione nelle aule del Parlamento.

pochi minuti per ricordarci che la democrazia, cioè il voto popolare e il giudizio del corpo elettorale su una legge o su una parte di essa, ossia appunto il *referendum*, devono avere regole certe e controlli certi. Questo decreto-legge va nella direzione di rendere attuabile la previsione di legge già esistente, che consente la raccolta elettronica delle firme di coloro che sostengono un *referendum*. ricordiamo i *referendum* storici del passato, ma sono proprio passati cinquant'anni e l'utilizzo di questo strumento dev'essere modernizzato e reso accessibile anche attraverso le nuove tecnologie. Il *referendum* è uno strumento fondamentale della democrazia, regolato puntualmente dall'articolo 75 della nostra Costituzione; si procede allo svolgimento del *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge (come già detto), quando lo richiedano 500.000 elettori o cinque Consigli regionali. Si tratta quindi di un numero di firme importante, che comporta un procedimento di raccolta, autenticazione e verifiche connesse. Dopo quel primo *referendum* proposto dalla Democrazia Cristiana, molte altre sono state le norme sottoposte al vaglio degli elettori. Le ricordiamo tutti, come ricordiamo le tante battaglie referendarie promosse dei Radicali. Cito solo i principali, per memoria: quello sul nucleare e quello sul finanziamento pubblico dei partiti, che hanno certamente condizionato le scelte successive altri, come a quello sulla responsabilità civile dei magistrati o a quello sull'abolizione di alcuni Ministeri, le scelte successive del Parlamento hanno dato invece un altro esito. Negli ultimi anni i *referendum*, il cui risultato, per essere valido, dev'essere comunque supportato dal *quorum* (maggioranza degli elettori e maggioranza dei voti espressi), hanno subìto successi e poi momenti di stanca. In ogni caso però questo istituto, previsto dalla Carta fondamentale e regolamentato dalla legge ordinaria del 1970, necessita di essere supportato da nuove forme di sottoscrizione. Siamo nell'epoca della firma digitale, della PEC e di una spinta sempre più pressante verso la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione. Quindi, per salvaguardare l'autorevolezza dell'istituto e dei controlli che lo regolano, viene rafforzato l'Ufficio centrale per il *referendum* del presidente della Corte di cassazione, per consentire le operazioni di verifica delle sottoscrizioni digitali; inoltre, deve diventare operativa la piattaforma digitale. Pur semplificata, l'attività di raccolta delle firme deve dare garanzie in termini di autenticità e semplificare l'attività di verifica. importante anche il fatto che ora venga introdotta la disciplina della piattaforma telematica per il *referendum*, per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* e le iniziative legislative popolari. modo è fondamentale, altrimenti non avrebbe senso, aver individuato una società di informatica per il completamento, la gestione e la manutenzione della piattaforma. Per queste ragioni, i senatori di Forza Italia voteranno a favore del decreto-legge

per le irragionevoli restrizioni nelle modalità di raccolta delle firme per la promozione dei *referendum*: moduli da compilare, firme, documenti, timbri e autenticatori rappresentavano un laccio che la burocrazia stringeva attorno al collo della partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica del Paese. Al fine di eliminare tale discrasia dell'ordinamento, il Parlamento aveva approvato in legge di bilancio - la legge n. 178 del 2020 - l'istituzione di una piattaforma di raccolta firme sui *referendum*, offrendo così la possibilità di abbattere qualsivoglia barriera rivolta all'attuazione di un pieno impegno civile e civico da parte dei cittadini. Purtroppo la normativa non è stata attuata e l'impegno è rimasto lettera morta. La piattaforma, che è stata introdotta con la legge che citavo prima, la n. 178 del 2020, articolo 1, comma 341, avrebbe dovuto essere attiva a gennaio 2022, poi è stata rimandata al 31 dicembre 2022 ed oggi si cerca di far fronte a questa sua ingiustificata inoperatività. Ricordiamo che agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita politica e alle scelte politiche del nostro Paese e dare concreta possibilità e facile attuazione al diritto costituzionale riconosciuto di promuovere *referendum* e leggi di iniziativa popolare dovrebbero essere il primo obiettivo di tutte le forze costituiscono un tema molto delicato, a cui il MoVimento 5 Stelle tiene particolarmente. Infatti, il MoVimento 5 Stelle ha più volte interpellato la Presidenza del Consiglio sulle ragioni di questo inspiegabile ritardo nell'adozione e nell'avvio di questo importante strumento di partecipazione alla vita democratica del Paese, ricevendo risposte rassicuranti, che poi si sono rilevate assolutamente non corrispondenti alla realtà dei fatti, vista la natura del provvedimento che ci accingiamo a votare. La disposizione transitoria che prevede la possibilità di raccogliere le firme necessarie per i *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione anche *online*, mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica, non è, allo stato, più sufficiente. Sappiamo bene che tale disposizione ha rappresentato un indubbio vantaggio ai fini della promozione dei *referendum* sulla cannabis e l'eutanasia legale, poi inusitatamente falcidiate dalla pronuncia della Consulta, ma dopo tre anni ci aspettiamo che finalmente venga dato seguito seguito a quanto stabilito dalla legge del 2020. C'è un problema: c'è una profonda differenza tra le due modalità. L'iniziativa transitoria, seppur lodevole negli intenti, non è gratuita, a differenza di quanto previsto per la piattaforma pubblica. Infatti, per mezzo di quanto disposto dalla normativa transitoria, il costo di ogni firma ricadrà sui comitati promotori. Un ostacolo economico all'attivazione della democrazia non da poco, considerato il fatto che, in caso di bocciatura, non è previsto alcun rimborso. Un motivo in più per considerare l'assenza della piattaforma pubblica un vero e proprio disincentivo a promuovere *referendum*. Sul punto si segnala anche che tale inerzia costringe le associazioni che propongono un *referendum* a utilizzare le piattaforme messe a disposizione dai privati. Allora una domanda ci viene naturale, quasi d'obbligo: perché i soggetti privati non hanno riscontrato tutti quei problemi che il Governo, invece, ha più volte sollevato quando è stato interpellato su questo gravissimo ritardo? Questa situazione, inoltre, ha creato un'intollerabile disparità, perché solo le associazioni dotate di ingenti risorse economiche possono rivolgersi ai privati e procedere speditamente con la raccolta delle firme attraverso l'uso degli strumenti digitali. Le associazioni più piccole e meno strutturate dal punto di vista economico purtroppo destinate quasi sempre a fallire nell'impresa di raggiungere il numero necessario per la proposizione dei *referendum*. Si tratta di un ritardo e di un'inerzia che per noi sono gravissimi, perché mettono a repentaglio la partecipazione democratica, fondamento della nostra impalcatura costituzionale. Riteniamo, viceversa, che il lavoro del Parlamento debba essere quello di migliorare sempre gli strumenti di partecipazione popolare e di democrazia diretta, perché la democrazia è sana quando moltiplica le occasioni di partecipazione e non certo quando le limita. Questo è anche uno strumento in più per porre un freno al calo della partecipazione che ormai si verifica ad ogni tornata elettorale. Dobbiamo e vogliamo invertire la rotta, restituendo credibilità alle Istituzioni e garantire, in maniera piena ed effettiva, la partecipazione dei cittadini alle scelte della vita del nostro Paese.

In ultimo, tenuto conto che il provvedimento in oggetto pone rimedio alla mancata operatività della piattaforma con un rafforzamento degli uffici della Cassazione, sul punto vorrei evidenziare e sottolineare che il MoVimento 5 Stelle, pur favorevole a detto rafforzamento, non condivide la scelta del Governo di ricorrere alla procedura dell'interpello, determina di conseguenza un depauperamento del personale di altre amministrazioni, poiché avrebbe invece preferito chiaramente il ricorso a nuove assunzioni. Signor Presidente, il nostro sarà un voto di astensione perché riteniamo che questo Governo non abbia fatto abbastanza e confidiamo che dietro questi continui rinvii e questi indugi ci siano solo l'inadeguatezza e l'impreparazione a cui purtroppo ormai ci ha abituato e non si celi piuttosto la malcelata volontà di limitare indirettamente la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del nostro Paese.

apparentemente sembrare anche molto tecnico e, in tal senso, ringrazio il relatore Zanettin per aver curato la questione e il dibattito in Commissione. Si tratta in realtà di un temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale del *referendum* per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni sulle richieste di *referendum*. Questo potrebbe magari anche annoiare chi ci segue, ma in realtà rappresenta una questione a monte che in realtà è molto interessante. Andiamo infatti anzitutto a sottolineare come si cerca e si cercherà sempre più di semplificare anche le procedure per la partecipazione della cittadinanza alla formazione delle leggi e al dibattito su di

cui finalità sono molto chiare e sono già state ricordate da tanti intervenuti. Si tratta di un provvedimento che cerca di adeguare il nostro ordinamento all'innovazione che è stata fatta fatta pochi anni fa con l'introduzione della raccolta delle firme *online* per l'indizione della richiesta di *referendum* abrogativi. Questo ha comportato una difficoltà nel lavoro di verifica delle firme da parte della Corte di cassazione e degli organismi deputati alla verifica delle firme. Il decreto-legge in esame serve a garantire alla Corte di cassazione di funzionare meglio in quest'attività di verifica, quindi con l'applicazione di personale aggiuntivo. Il decreto-legge in esame, però, finalmente introduce anche la piattaforma digitale per la raccolta delle firme *online* per la richiesta di *referendum* che dovrà servire in futuro

esame, pertanto, garantisce migliori condizioni per la verifica delle firme per l'indizione di *referendum* e quindi è certamente una normativa che aiuta a rivitalizzare un fondamentale strumento di democrazia diretta che è previsto in Costituzione e che, attraverso la raccolta delle firme *online,* ha certamente avuto un grande impulso. Altro poi sarebbe chiedersi - ma esula totalmente dal perimetro del decreto-legge come rivitalizzare un istituto che ultimamente ha zoppicato un po' anche per la scarsa partecipazione, ma questo sarebbe oggetto di una riflessione che va oltre il perimetro di questo provvedimento e che riguarderebbe invece qualche modifica costituzionale su cui varrebbe la pena anche di confrontarsi. Oggi però ci limitiamo a votare il decreto-legge in discussione, che aiuta a snellire il procedimento di raccolta e di verifica delle firme raccolte *online* per la richiesta di *referendum* e su questo noi siamo ovviamente d'accordo. È un provvedimento necessario e utile per rivitalizzare questo strumento importante di democrazia diretta. Signor Presidente, colleghi, come dice l'economista Brian Arthur, la tecnologia sta diventando organica e la natura sta diventando tecnologica.

Oggi l'epoca in cui viviamo ci impone un'accelerazione al fine di orientare e attualizzare gli strumenti che sostanziano la democrazia, come appunto le procedure di voto tramite i *referendum*.

e conoscenza, possono essere utili per rendere più rapida ed efficiente la risposta della pubblica amministrazione alle domande dei cittadini per rendere più snello il nostro ordinamento normativo. Siamo d'accordo sul fatto che il *referendum*, l'iniziativa legislativa popolare e la petizione rappresentano gli strumenti più alti di partecipazione diretta che i cittadini hanno per essere parte integrante del sistema

Il nostro partito, Fratelli d'Italia, per la sua storia, per la sua identità, ha sempre creduto nella partecipazione popolare alla vita democratica della Nazione; pertanto, a tutti quelli che puntano il dito asserendo falsità, dichiarando che noi di Fratelli d'Italia saremmo spaventati dalla partecipazione attiva attiva dei cittadini della politica, noi rispondiamo con i fatti, supplendo e colmando le mancanze precedenti. precedenti. Nel merito, il provvedimento in esame va proprio nella direzione di velocizzare e digitalizzare questo sistema, perché fino ad oggi le procedure che disciplinano i processi elettorali erano inadeguate. per far funzionare la piattaforma pubblica per la raccolta delle sottoscrizioni, prevista già dalla legge n. 78 del 2020, ma rimasta inattiva, si è ritenuto di incrementare il personale presso la Corte di cassazione. grazie a noi, si autorizza l'impiego in via temporanea di 100 lavoratori per smaltire il lavoro arretrato, ma soprattutto si rende operativa e all'avanguardia la gestione della piattaforma per offrire gli standard di sicurezza richiesti, quando si parla di una materia così sensibile che attiene alla democrazia.

ho sentito prima l'intervento - che avrebbe dovuto invece semplificare, non hanno snellito affatto le attività di verifica e nemmeno garantito la sicurezza dell'autenticità della raccolta delle firme. Ora, la piattaforma rimasta in fase di test diventa operativa attraverso un accordo già siglato nel maggio del 2023 tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e quello per la transizione digitale del Ministero della della giustizia, che completa le fasi di auto-attuazione della piattaforma e sancisce il passaggio della gestione al Ministero di giustizia (Mig). Quindi, dal nulla di fatto dei Governi precedenti alla risolutezza e serietà di Fratelli d'Italia, che rende concreti e attuabili gli strumenti per permettere la partecipazione democratica degli italiani.

viva il popolo italiano, che ad oggi ritorna a essere parte attiva della politica della Nazione.

sulla situazione di Alexei Navalny, come provo a fare di tanto in tanto, ma questa volta mi pare che sia particolarmente importante. Navalny non è apparso in uno dei videocollegamenti che avrebbe dovuto fare per rispondere alle molte accuse pretestuose che gli sono rivolte e non era apparso neanche in un collegamento del 7 dicembre. Le autorità russe dicono che ci sono stati problemi con la fornitura di elettricità. Gli avvocati di Navalny non hanno potuto vederlo, nonostante abbiano passato un giorno intero fuori dal carcere. Un mese fa i suoi tre principali legali sono stati dichiarati terroristi e arrestati, il che ha comportato la fuga dalla Russia degli altri legali e anche un segnale potente a tutti gli avvocati russi che chi prova a difendere Alexei Navalny è in pericolo. A Navalny sono negate le visite e le telefonate e le lettere sono bruciate dalla censura. Finora, per sapere che fosse vivo, potevamo soltanto avere la testimonianza degli avvocati che potevano incontrarlo davanti ai secondini e la sua apparizione nelle videoconferenze. In questo momento, non c'è più tale tipo di rassicurazione. Non sappiamo se sia vivo. Sappiamo che ultimamente era stato

ogni dieci giorni e stia continuando a perdere un peso enorme. Non si hanno notizie di lui. Una delle possibilità è che sia stato trasferito in un'altra prigione. Sono trasferimenti che durano un tempo incredibile, che non può essere misurato, e tutto questo avviene quando quando Vladimir Putin annuncia la sua ennesima candidatura alla presidenza della Russia. Allora, tramite lei, signor Presidente, vorrei chiedere al ministro Tajani - che oggi si è espresso sulla questione - di farsi vivo presso l'ambasciatore della Federazione Russa a Roma per esprimere la massima preoccupazione non solo del Governo italiano, ma dell'intero Parlamento. Noi abbiamo il nostro sguardo sulla sorte di Alexei Navalny e di tutti i dissidenti che si oppongono al regime di Putin e questo Putin deve saperlo. *(Applausi)*. L'ambasciatore russo faccia sapere al suo Governo che il Parlamento italiano è vigile, che non perderemo d'occhio questa situazione, che siamo qui presenti e che il mondo osserva quello che accade. I crimini contro i dissidenti russi e contro Navalny in particolare non accadono nel silenzio e non accadono lontano dallo sguardo di tutti noi.

Signor Presidente, sottoscrivo le parole del collega Scalfarotto. Per la verità non è la prima volta che quest'Assemblea richiama la situazione, a dir poco intollerabile, in cui versa Navalny, com'è capitato qualche settimana fa. È chiaro che noi come senatori siamo concentrati sulle questioni che riguardano il nostro Paese, ma l'Italia ha una tradizione antica di attenzione al rispetto dei diritti umani e certamente quello che sta capitando e che è capitato a Navalny non si addice a una democrazia, come non lo è più la Russia di Vladimir Putin. Purtroppo di questa persona non si hanno notizie e le poche che la stampa fa trapelare sono a dir poco inquietanti, non solo perché non si hanno più tracce di dove sia Navalny, ma perché addirittura il suo collegio di difesa - come ha sottolineato prima il collega Scalfarotto - è stato arrestato. Questa persona è stata sottoposta ad un carcere duro e ha perso molti chili. È evidente a tutti che si tratta di un oppositore di Vladimir Putin e di una persona che ha avuto il coraggio di denunciare ciò che da anni accade all'interno della Federazione Russa e io credo che un Paese come il nostro, una democrazia come l'Italia, non possa far finta non possa accettare che persone che provano ad affermare, all'interno della Federazione Russa, la validità, l'efficacia e la difesa dei diritti umani vengano sottoposte a queste torture, perché io non ho un un termine diverso per definire ciò a cui è stato sottoposto Navalny e quelli che come lui non accettano le angherie e le violazioni dei diritti di Vladimir Putin. Allora anch'io mi associo e come Azione lo facciamo tutti insieme - alla richiesta che è stata avanzata prima dal collega Scalfarotto, affinché il Governo e in particolare il Ministro degli affari chiedano, nelle sedi opportune, verità e chiarezza sullo stato di salute e sul luogo dove si trova Navalny. sappiamo che questa è una stagione difficile, in cui addirittura si mettono in discussione gli aiuti all'Ucraina. Noi non abbiamo dubbi che si debbano difendere l'Ucraina e il suo diritto ad esistere, così come si devono difendere Israele e l'Iran libero.

che riguardano il mondo e naturalmente siamo tutti tesi a costruire pace giusta, sia in Ucraina, sia in Medio Oriente, ad un certo punto arriva alla nostra attenzione, soprattutto in certi giorni e in certi momenti, la realtà di alcuni regimi. Il fatto che di Navalny, il dissidente, da giorni non si abbiano notizie, conferma quanto dispotico e quanto dittatoriale sia il regime di Putin, che mette in carcere e fa scomparire i suoi oppositori oppure usa o fa usare metodi per sbarazzarsi del tutto degli oppositori e così pure della stampa o dell'informazione che vogliono raccontare la verità di quel regime. Contemporaneamente, come ha rilevato il nostro collega, senatore Sensi, con un *tweet* fulminante, l'altro giorno angosciava vedere quella sedia vuota a Oslo, quando Narges Mohammadi, che giace nelle sanguinarie carceri del regime iraniano, non è potuta andare a ritirare il premio Nobel. C'erano solo i suoi familiari. Vogliamo dimenticare quello che accade in Bielorussia? No, non ci è consentito, quando le oppositrici del regime di Lukashenko, anche loro, sono incarcerate. Quello che voglio dire è che esistono ancora, e non sono soltanto questi, regimi per i quali la democrazia è il nemico. E noi sappiamo che, quando si muovono questi regimi, anche con le guerre, lo fanno non solo contro un popolo e contro un Paese, ma contro tutti noi. Infine, signor Presidente,

qualcosa da ricordare negli anniversari, ma dev'essere una pratica quotidiana. Pratica che ha dimenticato, poche ore fa, quel deputato dell'ultradestra del Parlamento polacco, il quale, dando una nuova prova di quanto l'antisemitismo in questi giorni e in questo periodo sia drammaticamente presente, ha avuto l'ardire di spegnere la Menorah, nel Parlamento polacco che ieri, per fortuna, ha conosciuto un cambio. Ci associamo alle parole che abbiamo ascoltato, Abbiamo veramente allargato il campo per dire che questi episodi non possono essere ignorati, ma debbono essere al centro del nostro impegno quotidiano.